anche in forma forfettaria, e voglio spiegare il perché di questa richiesta. La forma forfettaria per piccoli importi

relativamente alle spese di viaggio o a una colazione, e costringerli a fare una raccolta ossessiva di scontrini per poter giustificare tale piccolo rimborso mi sembra davvero una grande cattiveria.

Visto che nel disegno di legge c'è la volontà di fare una previsione di semplificazione, questo sarebbe davvero un esempio concreto. L'altro emendamento riguarda i centri di servizio. avuto direttamente questa esperienza per circa una decina d'anni in Toscana, e devo dire che il centro servizi per il volontariato toscano ha funzionato egregiamente,

a una semplice erogazione di denaro ma finanziava progetti. Si tratta di progetti innovativi, che hanno accresciuto la potenzialità e la capacità di progettazione delle associazioni.

con quel bando si era riscontrata una notevole crescita di queste associazioni. Chiediamo, quindi, di inserire soltanto la locuzione «in particolare» per non ridurre i centri di servizio a mere officine di formazione, che poi finisce per essere effettuata prevalentemente dalle strutture degli stessi centri di servizio; strutture che - queste sì - forse avrebbero avuto davvero bisogno di un ridimensionamento e di una riorganizzazione.

Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 5.273, che riguarda la lettera *f)* del comma 1, che prevede l'istituzione del consiglio nazionale del terzo settore come organismo unitario di consultazione degli enti del terzo settore. Giustamente, la lettera *f)* sottolinea l'importanza che questo consiglio valorizzi il ruolo delle reti associative; ma è molto importante che esso valorizzi anche la varietà delle tipologie di enti, in quanto diventerà un organo rappresentativo di questo settore e un organo di consultazione, richiamato anche in altri punti

Presidente, parliamo di terzo settore, del sociale, delle associazioni, delle cooperative, delle fondazioni. Vorrei illustrare il mio ordine del giorno G5.101, con il quale chiedo al Governo che si faccia finalmente giustizia e si cominci a riconoscere una figura che ad oggi in Italia non esiste, non è riconosciuta. È riconosciuta in Francia, in Spagna, in Gran Bretagna, in Romania, persino in Grecia; ma qui non se ne parla ancora. Pertanto, mi piacerebbe che il Governo

*(CoR)*. Signor Presidente, si stanno inseguendo agenzie di stampa che, usando il condizionale, informano che potrebbe esserci una cittadina italiana fra le 34 vittime di Bruxelles. Questo naturalmente determina un ulteriore motivo di angoscia in tutti noi e indubbiamente mi induce a chiedere, per il suo tramite, che il Governo, nei modi e nei tempi che riterrà (io spero con urgenza), venga a riferire all'Assemblea.

già previsto nell'articolo 4, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Agenzia delle entrate. È proprio su questo punto che si

cui si chiede al Governo che non si faccia *business* sull'emergenza; che non si facciano utili e guadagni sulla miseria e sulle disgrazie altrui;

impegna il Governo ad adottare misure utili a far sì che le cooperative sociali che ricevono finanziamenti pubblici nella gestione dell'emergenza migranti utilizzino l'intero ammontare delle risorse esclusivamente per tale finalità.

richiesta di poter estendere l'aliquota IVA agevolata alle associazioni che trasportano i disabili.

donazioni dal privato in maniera superiore a quanto avviene oggi. Sappiamo che le donazioni in Italia sono piuttosto rilevanti anche dal punto di vista quantitativo, mentre riteniamo che le risorse pubbliche nel campo dell'innovazione sociale

favorevole con la seguente riformulazione: sostituire le parole da: «la specificità» fino alla fine della lettera con le seguenti: «le tutele dello *status* di volontario e la specificità delle organizzazioni di volontariato ai sensi della legge n. 266 del 1991, incluse quelle operanti nella protezione civile».

«le tutele dello status di volontario e la specificità delle organizzazioni di volontariato ai sensi della legge 266/91, incluse quelle operanti nella protezione civile;».

il dispositivo di impegno venga sintetizzato nella seguente espressione: «A valutare l'opportunità di adottare disegni di legge recanti norme per il riconoscimento e il sostegno del *caregiver* familiare». Propongo infine

«le tutele dello status di volontario e la specificità delle organizzazioni di volontariato ai sensi della legge 266/91, incluse quelle operanti nella protezione civile;».

piccola modifica. Il senso dell'emendamento 5.206 è di tenere conto del fatto che, quando parliamo di persone che svolgono un lavoro volontario all'interno del terzo settore, questo può avvenire nell'ambito di associazioni di solo volontariato, come all'interno di associazioni miste in cui c'è anche chi svolge l'azione di volontariato. La proposta di emendamento e anche la riformulazione del relatore vanno in questa direzione. Chiederei però di porre attenzione sul punto specifico che riguarda chi opera come volontario e, più in generale, chi opera nelle attività di protezione civile. La riformulazione del relatore,

della specificità degli operatori di protezione civile, in quanto ricadano nell'ambito coperto dalla legge n. 266 del 1991 sulle organizzazioni di volontariato. Chiedo dunque che, all'interno di questa legge e in particolare all'interno della

dell'organizzazione della Protezione civile, pur non ricadendo nell'ambito della legge n. 266 del 1991. Credo che quel tipo di organizzazione meriti un'attenzione specifica e, quindi, chiederei al relatore la possibilità di un'ulteriore riformulazione dell'emendamento, che sostituisca la parola «incluse», con le parole «e

a quello successivo, identico al proprio. Evidentemente ci potrebbe essere una recondita intenzione di far decadere i subemendamenti all'emendamento 5.270, cosa che non trovo assolutamente corretta. Senatore D'Alì, lei ha preceduto puntualmente ciò che alla Presidenza non è sfuggito: è una riformulazione-resurrezione dell'emendamento

che non sono quelle del volontariato.

è giustificata dal fatto che anche ai volontari operanti e alle organizzazioni di volontariato

di una precisazione rispetto alle organizzazioni di Protezione civile nasce dal fatto che esse hanno, com'è noto, un regime e contratti anche pubblicistici, ma ciò non vuol dire che non ricadano nell'ambito della legge n. 266. In questo modo, dicendo che vale per tutti la specificità delle organizzazioni di volontariato, incluse quelle operanti nella Protezione civile, si dice che

L'ho detto con chiarezza cinque volte. È stato chiarissimo. Legga il Resoconto successivamente. Se era distratto, non ci posso fare niente. Era il subemendamento ed era chiarissimo ai colleghi. Ho anche citato i tre primi firmatari, nemmeno solo il primo. Lo ricordo a memoria. era in corso la votazione, senatore.

affinché, oltre a riconoscere il ruolo delle persone che lavorano e contribuiscono tantissimo al nostro *welfare* in silenzio,

totale condivisione della presa in carico e, prima ancora, della presa di coscienza dei problemi che patiscono le famiglie che hanno familiari in certe condizioni,

a queste famiglie sfortunate che necessitano di tutto l'aiuto possibile, sussidiario, ma anche dello Stato. *(Applausi della

per manifestare l'adesione del mio Gruppo all'ordine del giorno presentato dalla senatrice Bignami, il cui contenuto, che potrebbe sembrare estraneo all'oggetto proprio del provvedimento,

che l'Assemblea si impegni, con un voto sull'ordine del giorno, a coltivare detta questione, che non solo è centrale per la tenuta complessiva del nostro sistema di *welfare* e ricade esclusivamente - o quasi - sulle spalle di donne che spesso continuano anche a lavorare all'esterno, ma rappresenta anche un capitolo delicatissimo e molto impegnativo per la riconoscibilità di un sistema di *welfare,* come quello italiano, che sia adeguato a uno *standard* di stampo europeo.

«superamento del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale...» e poi più avanti, alla lettera *g),* di «previsione di requisiti uniformi per i registri e per gli Osservatori nazionali e regionali».

prima del voto sull'articolo 5, perché ci si renda conto anche di come queste leggi avranno difficoltà di attuazione solamente perché hanno delle contraddizioni interne.

un rimborso forfettario credo sia oggi un tema da rimettere in discussione. Magari sarebbe stato interessante affrontare seriamente la questione del contratto collettivo nazionale.

seguenti parole: «a valutare l'opportunità di avviare, attraverso la delega di cui al provvedimento in esame, una revisione della disciplina vigente in materia di cooperative sociali».

Sul volontariato e sull'associazionismo, sulla cooperazione sociale, sulle organizzazioni di promozione sociale e anche sull'impresa sociale abbiamo già legiferato in tempi recenti. Forse la più antica di queste legislazioni è quella sulla cooperazione sociale. Nel caso delle imprese sociali, la legge istitutiva risale al 2005, cioè a dieci anni fa.

Quindi, con questa delega specifica sulle imprese sociali noi deleghiamo il Governo a riordinare e a rivedere la disciplina. Ora, l'impresa sociale in Italia è stata ed è un *bluff*. L'impresa sociale è, nel nostro Paese,

una specie di mostro mitologico, in cui devono convivere due figure, quella dell'impresa e quella del sociale, cioè quella dell'impresa capitalistica e quella di un'impresa che, invece, ha caratteristiche sociali definite dall'articolo 1 del disegno di legge delega Perché l'impresa sociale è, quindi, un *bluff* e una leggenda metropolitana? In sostanza, o si remunera il capitale o non c'è una reale intenzione di intervenire, come impresa capitalistica, all'interno del terzo settore: i risultati ottenuti dal 2005 a oggi lo dimostrano.

Infatti, l'unica struttura societaria, l'unica società di capitali che può essere collocata

perché un'impresa, che deve o dovrebbe rimanere collocata solo nell'ambito del sociale, per funzionare ha bisogno di introdurre norme non leggere di stampo capitalistico, come la remunerazione del capitale, prevista,

«prevalentemente» significa che, rispetto al passato, mettiamo all'interno del terzo settore un società capitalistica, che può remunerare il capitale con un'attività sociale,

che il Parlamento debba, una volta per tutte, chiudere il capitolo davvero increscioso delle imprese sociali che - come ripeto - non sono né imprese, né sociali.

non ci sia solo un'ambiguità o che essa sia soltanto nelle parole, perché nelle intenzioni, che traspaiono chiaramente, si ravvede questo cedimento al mercato, in un settore che invece ha un'identità forte, soprattutto in Italia, rispetto a esperienze di altri Paesi. Abbiamo dedotto queste intenzioni dal rifiuto e dai pareri negativi dati su tutte le specificazioni che potevano vincolare maggiormente il Governo e garantire coerenza tra parole e fatti, parole e fatti, soprattutto quando i fatti, intendo dire i decreti legislativi, sono futuri, L'ho già detto sulle riforme costituzionali, e l'ho ripetuto in tante altre occasioni: noi dovremmo avere fiducia in qualcosa quando abbiamo motivo di dubitare. Perché dubitare? Perché non si limita il volume d'affari, non si limitano le retribuzioni, non si limita la possibilità di destinare utili a questa o quella funzione che non siano quelle strettamente sociali e non vediamo una spiegazione diversa. Se si vuole allora difendere l'onorabilità di un settore, si fa in modo che non possano accadere e non possano essere facilitate quelle distorsioni che abbiamo visto con Mafia Capitale. Infatti, laddove non si limita la retribuzione

di finanziare - ad esempio - la cattiva politica, di intervenire in fatti di corruttela e questo noi non lo possiamo permettere. Se allora i miglioramenti non sono se le precisazioni vengono rifiutate e se il buonsenso viene respinto noi dobbiamo purtroppo pensar male e pensare che è meglio non avere una legge che avere una cattiva legge. Per questo il Movimento 5 Stelle voterà a favore dell'emendamento soppressivo dell'articolo 6.

come appunto prevede questa legge delega al Governo, sono abbastanza comuni. Si risolve la questione con il concetto della prevalenza, ma è indubbio, come diceva il senatore Luigi Marino, che quando la promiscuità è orientata a due scopi del modello societario, cioè quello di natura capitalistica e quello di natura sociale, è molto complesso e complicato stabilire quale prevalga, se lo scopo capitalistico o quello sociale. Peraltro, riuscire a far emergere la prevalenza dello scopo sociale su quello

probabilmente ci sarebbe stata maggiore tranquillità da parte nostra nel votare a favore di una delega in questo settore e in questa materia. Mancando una delimitazione chiara, anch'io ritengo che tra una cattiva norma e una non norma sia preferibile quest'ultima.

in quella legge che, come abbiamo visto in questi anni, ha trovato difficile applicazione, non soltanto da parte dei soggetti che la dovevano recepire, ma anche da parte degli enti locali che poi la dovevano applicare, ad esempio per

Ci stupisce che oggi si sia non solo proseguita quella strada, ma si sia addirittura scelta la strada che volge lo sguardo oltre il sociale. In realtà, infatti, in tema di remunerazione del

bastare svolgere un'attività di carattere sociale, perché il tema, in questo caso, è il profitto, l'attività sociale, l'utilità sociale e il coinvolgimento dei soci. Questa era la distinzione fondamentale tra l'impresa sociale e le cooperative. Lo stesso emendamento del relatore, laddove prevede che l'attività sia legata, piuttosto che allo svolgimento delle attività statutarie, al conseguimento dell'oggetto sociale, ci fa capire che che l'intento della maggioranza e del Governo è quello di spostare l'attenzione proprio sul valore dell'impresa e, quindi, sul valore imprenditoriale. Per tutti questi motivi esprimiamo le nostre forti perplessità sull'articolo e voteremo a favore dell'emendamento del

sostenere la finalità sociale e solidaristica che sottende l'intero disegno di legge, quando, fin dall'inizio, promette un solido dei principi costituzionalmente protetti della sussidiarietà e della solidarietà, ma, di fatto, sembra non declinarli in modo puntuale e preciso, laddove il principio di di proporzionalità o, se vogliamo, il principio di prevalenza potrebbe, in qualche maniera, non garantirsi, agganciandosi anche a quanto previsto dall'articolo 9, con l'emendamento che è stato proposto dal che è stato proposto dal relatore. Questo è il motivo per il quale, in linea di principio, nutro le medesime perplessità e ritengo che uno dei punti di maggiore criticità dell'intero impianto di una legge necessaria

di Forza Italia - che adesso sono preoccupati della deriva imprenditoriale o capitalistica, che occorreva probabilmente mettere mano ad una legge - votata dai Governi di centrodestra - che, appunto, rivelava non pochi limiti, tant'è che praticamente non vi sono imprese sociali in Italia, se non in una Regione perché opportunamente incentivate. Sono almeno tre i limiti forti che la legge del 2006 contiene. Il primo è la totale impossibilità di distribuire alcun utile. Non è ragionevole pensare - come ha fatto il legislatore nel 2006 - che anche le imprese

esclude ogni tipo di agevolazione dal punto di vista dell'IVA e di altri vantaggi che, per esempio, il regime ONLUS consente, e che invece le imprese sociali non possono adottare. quindi messo mano - introducendo pienamente il concetto di impresa sociale dentro al terzo settore - a questi limiti, in primo luogo vincolando la possibilità, che viene introdotta, di remunerare il capitale esattamente nel limite - lo sottolineo - previsto per le cooperative a mutualità prevalente. Quindi, ciò che oggi è già consentito anche alle cooperative sociali, e cioè una modesta remunerazione eventuale del capitale investito - sostanzialmente per mantenere il valore reale del capitale - viene riconosciuto a tutte le imprese sociali - quindi anche Srl, SpA, e non solo alle cooperative - che vorranno scegliere questa formula. Non è un incentivo potente all'investimento di capitali, che vogliono tornare nel loro investimento ad essere redditizi, ma è certamente un modo per non escludere *a priori* che questi investimenti ci possano essere. una*partnership*, e quindi modelli gestionali dove anche i privati e la pubblica amministrazione possono entrare, seppure in quota minoritaria, dentro le imprese sociali. Pertanto, quel contenitore diventerà una proposta potente, nelle nostre intenzioni, per affrontare sfide complesse, come sono per esempio le ristrutturazioni di immobili, che poi vanno a gestione sociale, ed altre, dove probabilmente è necessaria anche una formula mista per affrontare, appunto, queste sfide così difficili. Il terzo vantaggio che viene inserito l'impresa sociale, in quanto pienamente collocata nell'alveo del terzo settore, beneficia delle stesse misure agevolative di tipo fiscale e di incentivo che sono previste già oggi per le cooperative sociali oppure per le associazioni e le fondazioni

che noi pensiamo possano essere meglio affrontate con lo spirito del terzo settore. Questa è la logica che ci ha portato ad una scelta anche molto equilibrata. Ricordo, per esempio, che, rispetto al testo della Camera, proprio in riferimento ai pericoli che anche il collega Endrizzi ha rappresentato, abbiamo eliminato quel riferimento per cui si consentiva una maggiore elasticità nella remunerazione del capitale con la formula «differenziabili anche in base alla forma giuridica» del soggetto che acquisiva la qualifica di impresa sociale. Abbiamo escluso questa possibilità e, quindi, il vincolo è per tutti quello della mutualità prevalente, che - secondo noi - è equilibrato e consente di eliminare sovrapprofitti che diversamente si sarebbero potuti prefigurare. È in questa logica che abbiamo pensato e ripensato al concetto d'impresa sociale, secondo noi aggiornandolo e rendendolo finalmente convincente e competitivo, pur dentro vincoli e limiti molto stringenti. vorrei argomentare al senatore Luigi Marino, il quale evidentemente, anche per le sue esperienze precedenti, conosce bene questo campo, che le sue argomentazioni sono contraddittorie. L'intento del Governo e della delega

normativa. Essa però introduceva nella qualifica d'impresa sociale un insieme di vincoli, opportunamente finalizzati a mantenere a mantenere la finalità sociale, ma nessuna possibilità per queste imprese di potersi effettivamente sviluppare come imprese sociali.

possa avere oggi anche altre forme giuridiche, con elementi di sostegno e facilitazione, in funzione però del vincolo sociale, cioè della prevalente destinazione degli utili che queste imprese realizzano. Tra l'altro, noi come Italia siamo stati antesignani della legge sulla cooperazione sociale negli anni Novanta ed abbiamo aperto una strada che poi in Europa si è diffusa.

nell'affrontare e risolvere una serie di bisogni e di servizi, che hanno bisogno anche di attori nuovi sul piano imprenditoriale.

nel senso che mette insieme l'esperienza delle cooperative sociali con quella delle imprese sociali, fa - com'è stato fatto in passato - un polpettone che condisce per il Parlamento. Sono cose completamente diverse. La contraddittorietà, su cui ha voluto incentrare il suo intervento il sottosegretario Bobba, è è nel fatto che non si può fare la quadratura del cerchio: o sta in un settore o sta in un altro settore. Cercare di trovare la figura mitologica che mette insieme un'impresa di stampo capitalistico e lucrativo con un'impresa che invece è soltanto vocata al sociale è una forzatura che si vuol fare solo in Italia. In Italia c'è chi vuol fare impresa con la cooperazione sociale; altrimenti si fa un'impresa capitalistica, che è sociale di per sé, perché un'impresa, una SpA è di per sé un'istituzione sociale, se produce reddito e ricchezza. Quindi, non c'è neanche bisogno del sociale, ma deve stare nelle regole capitalistiche; se viene nelle regole del terzo settore, fa il terzo

configurazione della presenza nel nostro ordinamento di imprese sociali, cooperative sociali, fondazioni sociali. Stiamo mettendo insieme una pericolosissima accozzaglia di iniziative che poi, trasferite al Governo per la delega, potrebbero generare addirittura punti franchi per dei modelli che hanno già dimostrato

i nobili intenti della socialità, si nascondono grosse e purtroppo dannosissime truffe ai danni dell'intera collettività nazionale. Ribadiamo pertanto il voto favorevole all'emendamento presentato dal

noi già viviamo in una Nazione in cui l'iniziativa privata è sottoposta al raggiungimento del fine sociale dell'impresa, che fu uno dei compromessi dei Padri costituenti, allorquando si scontrarono all'interno dell'Assemblea costituente coloro che erano di matrice socialista con coloro che erano di matrice liberale.

le partecipazioni statali e la *golden share*; cioè ha consentito sotto l'etichetta «sociale» le più grandi nefandezze anticapitalistiche, talché siamo ridotti in braghe di tela per l'enorme debito pubblico. Orbene, credo che ciò che è sociale

può maturare un vantaggio o una perdita. Ma questo è il fine dell'alea che corre l'imprenditore. Quando noi diamo l'appellativo di «sociale» a un'impresa, non possiamo trasformare qualcosa che non dovrebbe avere fini lucrativi, anche se ricordo agli astanti che il profitto non va confuso con i profittatori, ma è sacro come il salario.

di colui che si muove a intraprendere qualcosa, è una grande sciocchezza. Bisognerebbe però chiarire. Vi parlo del campo sanitario. Ci sono cosiddette cooperative sociali che hanno all'interno come soci le mogli di eminenti politici o di consiglieri regionali, che dividono gli utili e godono di linee di privilegio e di vantaggio rispetto agli imprenditori lucrativi. Adesso cosa vogliamo fare? Vogliamo dare loro un altro vantaggio? Non solo hanno i vantaggi dovuti alla cosiddetta socialità; adesso volete trasformarli in qualcosa che li faccia somigliare di più alle imprese? Allora, togliete i vantaggi perché la competizione si può sviluppare a parità di regole. Se voi all'impresa sociale volete conferire altre caratteristiche, come Marino giustamente ha detto, state facendo una truffa: state favorendo determinate tipologie d'impresa

Se non ci fosse stato un comune sentire, compreso tra le file del Partito Democratico, su un argomento come questo, avremmo votato. Se il Sottosegretario non avesse contato uno a uno i suoi voti, non avrebbe chiesto l'accantonamento. Ma su questi temi è possibile che non si riesca a lavorare in maniera seria senza arroganza, onorevole Sottosegretario? La risposta del sottosegretario è stata uno schiaffo a questo Parlamento e non l'ha fatto verso l'opposizione, ma verso persone che hanno una storia personale che hanno messo a disposizione facendo politica. Un po' di umiltà qualche volta serve. Non ci si deve sentire sfregiati se, ogni tanto, si dice sì a un emendamento di buonsenso. Adesso accantonate; votiamolo invece! Abbiate la forza di mettere la stessa arroganza con il pulsante e schiacciare contro l'opinione di tutto questo Parlamento. Abbiate questo coraggio.

È già intervenuto

conseguente alla richiesta di accantonamento del Sottosegretario indubbiamente non è un atto, così come è stato definito, di arroganza e prepotenza; anzi, anzi, devo dire che, se un rappresentante del Governo, dopo aver ascoltato i rilievi e le osservazioni

si ferma un attimo a riflettere sulla decisione che deve esprimere, a me pare un gesto di umiltà e saggezza.

sta succedendo di tutto e di più a livello internazionale. Pertanto, che i Governi e i Parlamenti si abbraccino e cerchino di trovare delle soluzioni più ampiamente condivise è una cultura che non posso

In ogni caso, ho accolto con favore la richiesta di accantonamento avanzata dal Governo, perché finalmente si esce definitivamente allo scoperto sul piano politico in quest'Aula.

era già previsto all'articolo 4, che è stato votato, come si può evincere dalla documentazione.

il potenziale stralcio dell'articolo 6, che adesso dobbiamo mettere in conto, va a impattare anche su norme già votate.

si definisce l'impresa sociale in base alle finalità definite dall'articolo 1, nel quale però si esplicitava anche che quelle finalità erano esercitate senza fini di lucro;

che poi a questo punto sta diventando certezza, viste le resistenze e la trincea che si sta scavando. Mi riferisco cioè al fatto che nel provvedimento in esame, come un cavallo di Troia, si sta infilando lo smottamento dalla gratuità al lucro, attraverso modalità che consentiranno

fare chiarezza una volta per tutte. Chiedo pertanto di non procedere nell'esame e di decidere ora una pausa per arrivare a una

dell'esame si vedrà, tanto che ho detto di votare gli emendamenti e di tenere in sospeso la votazione dell'articolo. Mi sembra un modo ragionevole di procedere e che quindi non escluda le conseguenze perché, anche se fosse bocciato l'articolo 6, ci sarebbero riferimenti su parti già votate, e quindi non possiamo

ma credo che sia il momento di una diversa valutazione, non su questo provvedimento ma sullo stato attuale di questa maggioranza.

ancora quella capacità di legiferare che non avrebbe se non ci fossero nuove componenti che hanno aderito in maniera ormai omogenea alla maggioranza. Credo che ormai la riunione dei Capigruppo di maggioranza si sia estesa a sei o sette componenti quando c'è da decidere cosa fare.

cari colleghi e care colleghe, voi state prendendo in giro la gente. Lo dico dall'ala più sinistra della destra e dall'ala di destra più a sinistra. Lo chiedo per i colleghi del Partito Democratico, che si stanno domandando, anche con un certa ansia, con chi ansia, con chi governano. Lo chiedo, in maniera molto semplice, da parlamentare, perché non è vero, signor Presidente, che la presenza in maggioranza si esercita unicamente avendo Sottosegretari o Ministri. Si esercita anche con degli interessi collaterali, legittimi, di rappresentanze che non sono necessariamente parlamentari. Vogliamo un passaggio parlamentare.

Ma la discussione che si sta sviluppando qui dentro è essenzialmente generata da questo ossimoro: impresa sociale.

definire un'impresa sociale lascia molte perplessità. Il collega Endrizzi, che oggi si pone il problema di separare il grano dal loglio, cioè quello che non ha scopo di lucro da quello che lo ha,

si invocano i principi di solidarietà politica, che non so cosa significhino, di solidarietà economica e di solidarietà sociale. La verità è che l'impresa è l'impresa. Il capitalismo e il mercato di concorrenza non lo cambiano né il Senato della Repubblica italiana e neanche le Nazioni Unite. le loro regole, che si basano sulla legge della domanda e dell'offerta e sul sistema dei prezzi, che sono basati sul gradimento degli utenti. Quello che è definito sociale dovrebbe essere spogliato del tutto dalle caratteristiche dell'impresa. Il senatore Endrizzi si meraviglia che sarà il Governo a fare l'elenco di chi può fare cosa,

È chiaro che, nel momento in cui si eliminano le regole del mercato e della concorrenza, è lo Stato che la fa da padrone. E lo Stato è di proprietà, o è governato, da chi, in quel momento, ha vinto le elezioni.

Presidente, vorrei tornare al punto vero, di merito, della discussione che si è sviluppata in Assemblea e che si è originata dall'emendamento soppressivo dell'articolo 6, presentato del collega senatore

di una domanda un po' fuori tempo, nel senso che, come ricordava il sottosegretario Bobba, già dieci anni fa, nel 2006 - peraltro con una legislazione giudicata assai avanzata in ambito europeo, tanto da diventare un modello per per successive elaborazioni culturali - si è deciso che l'impresa sociale andasse a buon titolo considerata nel campo del terzo settore. Questa scelta, operata prima alla Camera dei deputati e poi al Senato, seguendo una scelta politica compiuta dieci anni fa in questo Paese, non è mai stata messa in discussione durante i nostri lavori.

Vorrei anche aggiungere che il testo dell'articolo 6, rispetto a quello della Camera dei deputati, è assai più definito e assai più garantista di quelle che, ad esempio, poc'anzi il collega D'Anna ha considerato come finalità che - a suo senatore Lepri, peraltro in un rapporto

colleghi e molto puntuale per quanto riguarda la definizione dell'attività dell' impresa sociale, collocabile a pieno titolo nel settore più ampio, che è quello denominato come terzo settore. Ho quindi il sospetto - lasciatemi dire, colleghi, anche per il tono e i contenuti di molti degli interventi che si sono succeduti da quei banchi, in quest'ultimo momento

Ora, francamente, io mi permetto di dire che di tratta peraltro di un settore molto importante, anche

e di straordinario rilievo, non solo sotto il profilo del capitale economico, ma della qualità e della quantità del capitale sociale che vive, opera e produce in questo Paese.

- com'è normale in un'Aula parlamentare, di mera strumentalità politica una decisione che peraltro all'articolo 4 avete già asseverato, perché che l'impresa sociale stia nel terzo settore l'avete già stabilito con il voto sull'articolo 4. Io non ho niente in contrario, anzi, che si accantoni la votazione dell'articolo 6, che si rimediti questo testo, che i colleghi tornino su di esso a ragionare e a riflettere, ma per favore non parliamo d'altro. Quest'Aula ha già deciso che l'impresa sociale sta nel terzo settore. Se il testo proposto dalla Commissione e redatto con attenzione dal collega Lepri non viene considerato un testo soddisfacente, si valuteranno gli emendamenti ma non possiamo tornare a rimettere in discussione una questione strutturale. Lo dico perché talvolta si mette in gioco, per ragioni ovvie di opposizione e di strumentalità politica, un bene che sovrabbonda per importanza, per serietà e per qualità quella che può essere una polemica di giornata.

che abbiamo dimostrato, come molti altri colleghi dell'opposizione, di aver dato il nostro contributo, sia nel lavoro di Commissione che in quello dell'Assemblea.

per mettere tutti i colleghi, anche quelli che in Commissione non hanno seguito i provvedimenti, in grado di intervenire quando si accende la luce su questioni di particolare importanza, come ha fatto il senatore Marino. Il fatto, poi, che vi sia una legislazione in materia o che ne abbiano già parlato la Camera o la Commissione

Roma. Uno dirà che la colpa è stata della destra, un altro dirà che è stata della sinistra, un altro che è stato il sindaco Tizio, un altro che è stato il sindaco Caio; ma che l'opinione pubblica si sia preoccupata della gestione di

con finalità di interesse generale, destini i propri utili «prevalentemente» al raggiungimento degli obiettivi sociali, che a casa mia significa che il 49 per cento degli utili possono essere, invece, come in una società capitalistica, dati agli amministratori o divisi tra chi remunera il capitale. Pertanto, nel momento in cui sul pregresso che ha preoccupato tutta l'Italia si solleva un problema così serio,

La contraddizione è talmente gigantesca e palese che dopo non si può più dire che quello che è successo a Roma è colpa della destra o della sinistra: sarebbe colpa del Parlamento se non regolarizzasse in qualche modo una realtà che, per le caratteristiche spurie in cui si presenta, si sa già che determinerà

Presidente, faccio una riflessione sotto il profilo politico. Se io, parlamentare, all'interno di quest'Aula, dovessi esprimere un voto, ad esempio sull'articolo 4,

proseguendo nei lavori, sull'articolo 6 si aprisse un dibattito e una discussione e i colleghi all'interno del Parlamento, a prescindere che siano a destra o a sinistra, con grande tranquillità e serenità, nell'interesse del Paese, mi facessero rilevare che quell'atteggiamento che ho assunto e quel voto sono stati sbagliati e io allora prendessi una posizione e correggessi il mio percorso, nell'interesse della collettività e del Paese,

prendo una posizione completamente diversa e dico: «Attenzione, fermiamoci, accantoniamo; quell'articolo deve essere profondamente modificato, perché la sua applicazione potrebbe danneggiare gli interessi della collettività e del Paese»? Questa è la riflessione che faccio ad alta voce. Perciò non capisco come esperti di politica, personaggi presenti all'interno di quest'Aula da vent'anni, cerchino di additare, di responsabilizzare quei parlamentari che hanno assunto un certo atteggiamento, si sono accorti di avere sbagliato e vogliono correggere il proprio percorso, dicendogli indirettamente che si comportano male e che, siccome avevano scelto di approvare l'articolo 4, devono continuare a perseverare nell'errore, continuare a sbagliare, comportandosi

con un titolo che non vado qui a ricordare, fra coloro che sono presenti in quest'Assemblea parlamentare. È chiaro che la comune esperienza ci insegna di migliaia di emendamenti, indipendentemente da chi governa e da chi è

il dibattito che ha preceduto l'inizio dell'esame degli emendamenti all'articolo 7 ci lascia assolutamente sereni, ma vorrei dire anche indifferenti alle considerazioni fatte dalla presidente Finocchiaro. La verità è che La verità è che con l'articolo 6 - evitando le funzioni ispettive, come prevede questo emendamento all'articolo 7, anche su quelle che poi dovessero essere, ove mai si approvi l'articolo 6, le cosiddette imprese sociali - si vogliono introdurre degli elementi di enorme lesione del mercato, della libertà e della concorrenza, perché si tratta di imprese

quali punti di discriminazione porrà il Governo tra chi lavora nel privato e chi lavora nel cosiddetto sociale. Si potrebbero avere differenze fiscali, ma si potrebbero avere addirittura differenze in ordine alle graduatorie negli appalti nell'aggiudicazione delle forniture. Basta avere la possibilità o la fortuna - chiamiamola fortuna e non in modo diverso - di essere inseriti nell'elenco delle imprese sociali per poter avere dei vantaggi competitivi.

nella nostra legislazione una possibile discriminazione tra due imprese che fanno le stesse cose, ma una sotto il chiaro e trasparente regime di impresa economica - chiamiamola così, anche se c'è una certa sovrapposizione di termini, perché l'impresa è di per sé economia - e l'altra, invece, sotto il mantello della qualifica di impresa sociale, godendo in tal modo di tutta una serie di vantaggi. Ha perfettamente ragione il senatore Marino: questa previsione va eliminata, perché dobbiamo smetterla di entrare a piedi uniti nella libertà di concorrenza, di mercato e di autodeterminazione dei processi imprenditoriali,

la norma finale alle decisioni governative. Sappiamo poi cosa succede quando arrivano i decreti legislativi e quando anche la stessa maggioranza ritiene, nelle Commissioni, che il Governo esageri nell'esercizio della delega; sappiamo che non valgono questioni di costituzionalità e che non valgono pareri condizionati, perché poi il Governo tira dritto per la sua strada, secondo quello che gli conviene e che ha deciso. Quindi, approvando questo emendamento di ulteriore incisività sulle facoltà ispettive

la situazione in cui siamo, tuttavia voteremo contro questo emendamento, perché già il resto del provvedimento appesantisce sufficientemente un settore che dovrebbe essere caratterizzato dalla gratuità e dal mettersi al servizio degli altri.

con evidenti costi (dettagliati e coperti, come certificato dalla Commissione bilancio), direi che abbiamo una contraddizione in termini. Pertanto, voteremo contro questo emendamento.

Trovo assolutamente singolare che il Governo e l'Assemblea continuino a votare un testo che prevede che l'attività di controllo sulle possibilità sulle possibilità che un'impresa economica possa usufruire del titolo di «sociale» per poter avere degli evidenti vantaggi in termini di concorrenza

del controllo delle stesse da parte di chi le definisce e valutazione degli eventuali scantonamenti da queste regole sempre da parte di chi le ha definite

dei punti di controllo al di fuori di questo meccanismo a me sembra la soluzione più logica. In questo caso, la proposta del senatore Consiglio è che intervengano le Regioni a dare una valutazione. Può anche non essere

Presidente, io però volevo intervenire per una brevissima dichiarazione di voto sull'emendamento precedente dichiarandomi molto sorpreso che questo Governo, che pare abbia trovato nell'ANAC la fonte di tutta la saggezza e la verità, la voglia poi escludere dalle attività di controllo sulle imprese sociali. Quindi, questo mi rafforza nell'idea che il Governo in carica non vuole che sulle imprese sociali ci possano essere entità, al di fuori della sua stretta sua stretta cerchia decisionale, che possano eventualmente sollevare attenzione.

Presidente, l'emendamento del senatore Galimberti interviene sulle preoccupazioni che abbiamo già espresso e ribadiamo in questa sede. chiaro che la preoccupazione del mondo dell'impresa e del lavoro è che possano essere violate in maniera legittima (ossia in modo coerente con la normativa, ma non certo legittimo dal punto di vista delle regole che dovrebbero presiedere le forme

e continuo di queste attività, se non si vogliono mettere in dubbio le regole della libertà e della trasparenza nel nostro Paese e se vogliamo evitare

che siamo nel mezzo di un passaggio epocale importantissimo. La crisi economica, ma anche le nuove opportunità che tentiamo di mettere in campo per combattere la crisi economica, ci spingono a guardare con attenzione e profondità di pensiero e prospettiva

hanno accompagnato il sostegno alle famiglie, l'attività sussidiaria dello Stato e, in molti casi (come, ad esempio, quello della cooperazione bancaria) il sostegno all'economia reale. Mi riferisco a quell'economia che non entra nei santuari della finanza, quell'economia piccola e minuta che ha accompagnato lo sviluppo delle nostre famiglie e delle nostre imprese (perché per noi l'impresa e la famiglia sono in molti casi una cosa sola).

tra di esse vi siano anche quelle che non operano in maniera trasparente e pulita, godendo dei vantaggi competitivi che giustamente il senatore D'Anna sottolineava,

che gestisce i rifiuti, ma a una società a capitale misto pubblico e privato, perché non può perseguire in maniera coerente il *business*, il profitto e il miglior servizio al minor costo per i cittadini. Ciò detto, in questo caso stiamo parlando di attività sociali di tutela dei dritti civili e sociali, di promozione della partecipazione. Pertanto, nell'ipotesi che vi sia

che un cittadino veda frustrato il senso civico della denuncia. Il Governo non vuole controllare; lo lasci fare ai cittadini e almeno abbia il pudore di sostenerli. Invece, anche su questo emendamento è stato espresso parere contrario. Chiedo all'Assemblea, a questo punto, di assumersi una responsabilità. Il suo predecessore nelle funzioni di Presidente ha stabilito che potevamo procedere senza sapere bene se le imprese sociali erano incluse o meno. A questo punto, dobbiamo ritenere che lo siano, perché questa era la *ratio* del provvedimento. L'articolo 6 era - ed è

Signora Presidente, non possiamo votare a favore di questo emendamento, perché il concetto della denuncia anonima è assolutamente estraneo alla nostra cultura. Se un cittadino ha qualcosa da rilevare, deve farlo in assoluta chiarezza e assumendosi la responsabilità di ciò che fa. Non possiamo non evidenziare

omettere di fare controlli diretti, ma addirittura l'autocontrollo è riservato alle stesse imprese. Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un sistema disegnato

la pensiamo così. Ma è anche vero che è inconcepibile che esistano forme di autocontrollo in una materia sulla quale è stato affermato, anche dagli stessi esponenti della maggioranza, che, data la delicatezza della questione,

Senatore Marton, come ha visto, ho più volte richiamato la senatrice Fucksia al tema e non sono autorizzata a togliere la voce, perché questa è un'Assemblea libera, in cui si devono rispettare le regole.

regolare determinate norme nell'ambito della sua azione. Questo «anche», contenuto nel testo, resta indeterminato.

di dare al Governo deleghe del tutto indeterminate - e ce ne sono parecchie in questo provvedimento - oltre a non essere condivisibile, è soprattutto contro la Costituzione, la quale stabilisce in modo molto chiaro stabilisce in modo molto chiaro che il Governo può diventare legislatore solo sulla base di criteri precisi che definiscano non l'oggetto ma, per l'appunto, il criterio perché l'oggetto è insito nella cosa stessa. Quando si parla di criteri non si intende: diamo mandato al Governo di fare quello che gli pare in questo campo.

il mezzo migliore per conseguire i fini che si propone questo comma: non «anche» è quel mezzo. Se il Governo vuol fare qualcos'altro si scomodi a presentare emendamenti in cui viene autorizzato a fare altro, altrimenti abbiamo un altro incarico indefinito al Governo, Governo, che poi non rende conto neanche in casi straordinari e macroscopici del suo operato quando

altrimenti contravveniamo al principio della separazione dei poteri e, in altre parole, non siamo più una democrazia né uno Stato di diritto.

in gran parte utilizzano finanziamenti pubblici. Quindi, credo che l'inserimento di uno specifico riferimento al finanziamento pubblico sia assolutamente congruo.

della maggioranza nei confronti di forme di approfondimento dei controlli e dei rendiconti alimenta il sospetto, che noi abbiamo, che dietro questi meccanismi si possano configurare - come ho detto in altro momento - situazioni Non comprendo perché la maggioranza si rifiuti ostinatamente di approvare proposte di approfondimento di controllo

perché finalmente abbiamo qualcuno che collabora con noi in uno sforzo che finora abbiamo compiuto da soli. Mi spiace osservare che non abbia rilevato l'assenza dei senatori Augello e Aracri

il Governo deve dire da che parte sta. In qualsiasi modo siano erogati, che si tratti di appalti o di finanziamento dell'attività in quanto sussidiaria, attraverso le pubbliche amministrazioni, i

Vorrei che, da questo punto di vista, avessimo un chiarimento dal Governo: se veramente ritiene di poter scorporare o non finanziare o differire la responsabilità di controllo, nel momento in cui fatti gravissimi di corruttela si sono verificati qui a Roma, dove il soggetto politico responsabile e coinvolto era proprio il Partito Democratico. Credo sarebbe utile per tutti sgombrare questo dubbio. tutelare, proteggere, incentivare, valorizzare il patrimonio di iniziativa dei tanti cittadini italiani, prioritariamente non permettendo a una piccola minoranza d'infangare l'onorabilità di tutti.

Ora, sappiamo che le convenzioni bene o male recano criteri uniformi, a cui tutti si devono uniformare, e questi devono essere alla base del riconoscimento dell'attività.

daranno l'accreditamento a qualcuno piuttosto che ad altri, senza il quadro delle convenzioni che stabiliscono le regole per cui si può chiedere ed ottenere questo accreditamento. Il relatore introduce quindi un ulteriore elemento di fumosità,

di iniziative che possono godere dei vantaggi derivanti da questa norma. Già ritenevamo il testo, di per sé, opinabile, ma adesso a maggior ragione. Per questo il subemendamento 7.228/9, della senatrice Granaiola, che cercava di riportare al testo originario, sarebbe stato da accogliere, e spero che anche la maggioranza a questo punto voglia bocciare l'emendamento del relatore e quantomeno mantenere il testo originario,

io stesso ho scritto «ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6» - che non c'era alcuna pregiudiziale aprioristica rispetto alla presenza di alcune imprese sociali. Non è la stessa cosa parlare, ad esempio, di una cooperativa sociale di tipo A o di tipo B e in determinate condizioni, secondo determinate garanzie e secondo

Ma, nel momento in cui non vengono fatti salvi dei principi fondamentali e non ci può essere quella collaborazione a un utile miglioramento del testo, anche nella fase d'Assemblea, allora ci si pone il problema se, di fronte al muro e alla blindatura del testo, tutto il lavoro che stiamo facendo sia ancora utile e se sia utile quello fatto in Commissione. Infatti sono due le fasi previste ma, se nulla viene accolto delle indicazioni, allora la minoranza può ritenere che nessuna legge sia meglio che una cattiva legge. Nello specifico, poi, si ritiene semplicemente che una funzione di controllo non possa non essere finanziata. Ne ho parlato prima a proposito della sanatoria Boccadutri, ma vale anche in questo caso. Mi spiace che ci sia una bocciatura da parte della Commissione bilancio, nel momento in cui tante altre parti del testo, propugnate dal relatore e dal Governo, avevano chiaramente dei costi. Se noi Se noi rinunciamo a finanziare il controllo, legalità e onestà sono concetti vuoti.

potrà essere operata in sede di coordinamento del testo. Quindi, l'articolo 7 credo possa essere messo in votazione. È una questione di coordinamento e consequenzialità: non possiamo riaprire l'emendabilità dell'articolo 7,

Il presidente Gasparri - non in quanto senatore, ma in quanto Presidente - aveva detto in maniera chiara che si sarebbero votati gli emendamenti, ma non gli articoli. Se dobbiamo cambiare le carte in tavola dopo che

Colleghi, per rispetto al senatore Gasparri e alla Presidenza, sospendo la votazione dell'articolo 7, ma solo sull'articolo 7 e non sui successivi, perché non credo, laddove ci siano dei problemi di coordinamento del testo, si debba sospendere la votazione di un articolo, una volta votati gli emendamenti. Quindi, se questo era stato deciso prima, mi attengo alla decisione su cui fa conto l'Assemblea e sospendo la votazione finale dell'articolo 7 fino a quando sarà stata risolta la questione la questione dell'articolo 6. Procediamo al voto degli emendamenti sull'articolo 8, fermo restando che non è che dovunque ci sia un riferimento all'articolo 6 si possa non votare. Eventualmente, qualora l'articolo 7 venisse soppresso o modificato, in sede di coordinamento del testo, con una votazione dell'Assemblea (perché il coordinamento non sarà solo formale) verrà raccordato il testo degli emendamenti alla modifica intervenuta all'articolo 6.

l'attività di coordinamento serve a risolvere piccoli dettagli, e non a postulare una volontà politica di un'intera Assemblea. Assemblea. Non vedo come si possa desumere che il voto sarebbe stato favorevole o contrario... PRESIDENTE. Mi scusi, ma abbiamo già detto che non si voterà l'articolo 7.

l'ipotesi che nessuno sia contrario. Io sono contrario e lo dichiaro. Non è possibile postulare la volontà non solo di un Gruppo parlamentare come il Movimento 5 Stelle, ma dell'intera camera del Senato in base a quel che si deciderà dopo per quel che è stato votato prima. Credo che non ci si potrà limitare ad una mera attività di coordinamento perché, l'ho detto in dichiarazione di voto in più di un'occasione, l'inclusione o meno delle imprese sociali

di rinviare a mercoledì, ad un momento in cui si siano superate questioni di natura politica che insistono su un testo sul quale i Gruppi in Parlamento hanno più volte reiterato la propria disponibilità a trovare delle convergenze oggettive. Nel momento in cui lasciamo appese questioni politiche rilevanti, come quella posta dal senatore Marino, non facciamo altro che metterci nell'ottica di produrre un testo realmente non utile allo scopo che la proposta di norma si è prefissa. prefissa. Vorrei che verificasse se c'è la disponibilità dei Gruppi a rinviare ad un momento in cui il voto possa essere coerente con le soluzioni trovate Senatore, la valutazione della Presidenza è che si è disposto l'accantonamento di un articolo e questo non condiziona l'*iter* successivo. Era stata chiesta la sospensione della votazione dell'articolo 7 ed è stata data. Ora procediamo secondo la sequenza logica

Mi spiace dover recuperare la memoria della precedente gestione della Presidenza, ma l'accantonamento dell'articolo 6 è stato fatto su richiesta del Governo. Vorrei quindi sapere se il Governo ha sciolto le perplessità in ordine all'articolo 6 che lo avevano spinto a chiedere l'accantonamento e se il Governo pensa di poter procedere, prima di poter decidere se essere favorevole o meno all'accantonamento. C'era anche stato un voto dell'Assemblea

La differenza è che il suo Gruppo ritiene che non si possa e non si debba, mentre si può

che la Presidenza può decidere autonomamente sull'ordine delle votazioni. Ciò detto, siccome c'è stato un espresso voto dell'Assemblea, affinché la stessa sia confortata

un momento di decantazione rispetto al tema in esame. Prendiamo atto del fatto che, rispetto al Governo, il tempo è stato sufficiente. Abbiamo necessità di concludere l'esame dell'articolo 6 per approvare l'articolo 7, quindi siamo assolutamente a favore della proposta e auspichiamo che lo si faccia con celerità.

Debbo quindi capire che questo differimento è servito, non per far decantare l'Assemblea dai suoi bollenti spiriti, ma per far affluire un numero di voti utili o per convincere qualcuno che si era espresso a favore dell'emendamento 6.200, per cui, una volta fatti i conti, si può riprendere la

privato di una parte che, condivisibile o meno, comunque in sede di esercizio di delega può essere migliorata.

che voglio dire, perché lo penso e ad onore di verità. Il testo approvato dalla Commissione, ad opera dei commissari e del relatore,

Le mie obiezioni erano però di altra natura ed erano obiezioni di fondo e, nonostante l'invito, pur comprendendo la decisione del Capogruppo e del Gruppo di cui mi onoro di fare parte e che naturalmente impegna soltanto il sottoscritto, non posso, per gli argomenti che ho citato nei miei interventi, ritirare l'emendamento.

ovviamente rispondere al senatore D'Anna. Detto questo, credo che l'emendamento del senatore Luigi Marino sottenda una scelta di fondo, perché sospettiamo che attraverso questa legge non si voglia migliorare la vita del terzo settore, ma ci si voglia appropriare, con strumenti che spunteranno come funghi, anche del terzo settore.

perché nell'articolo 4 si stabilisce che tutti quelli che operano nel terzo settore sono uguali, e quindi sono sottoposti a determinate regole e vincoli, ma nell'articolo 6, se non passa l'emendamento del senatore Luigi Marino, si stabilisce che tutti sono uguali salvo coloro che possono godere di una posizione di privilegio rispetto agli altri, remunerando il capitale pagando adeguatamente i consiglieri d'amministrazione,

imponendo gli interessi propri o di un gruppo ristretto e difendendo a oltranza i propri amici, a danno di altre persone». Esattamente quello che voi state facendo con questo articolo 6 che è di tipo mafioso, in senso lato. Senatore Giovanardi, non credo possano essere qualificate posizioni politico-parlamentari su singoli emendamenti in questi termini.

si è sviluppato un dibattito abbastanza intenso ed un confronto che ho visto fortemente orientato al recupero del cosiddetto principio di buon senso, che tuttavia vedo completamente dissolto nel breve volgere di un'ora, né mi sembra che siano intervenuti elementi significativi tali da recuperare il principio della validità delle obiezioni che sono state mosse. che si è sforzato, con lodevole impegno ma con infruttuoso risultato, di spiegare gli effetti del vincolo della mutualità prevalente che sarebbero, a suo avviso, insiti nell'ambito dell'articolo 6; ma questo sembra, a parere dei più che sono intervenuti, assolutamente insufficiente. Infatti quando il sottosegretario Bobba ha accolto la richiesta di una di una riflessione e di un approfondimento, speravo che potesse esserci un passo in avanti nella direzione di sgombrare il campo da quelli che non sono più solo equivoci o interpretazioni artificiose o strumentali ma che sono effettivamente punti di gravissima vulnerabilità contenuti nell'articolo 6, con l'assoluta debolezza del principio di prevalenza a sostegno del valore di sussidiarietà e di solidarietà che innerva il provvedimento e di cui l'articolo 6 è la pietra fondamentale. Queste motivazioni provocano una condizione di grande delusione, per un verso, e purtroppo il rammarico nel dovere annunziare il voto favorevole all'emendamento 6.200, non mancando di osservare come e quanto il senatore Luigi Marino sia sempre uguale e se stesso, una persona che evidentemente della coerenza ha fatto la ragione della sua vita e di questo mi rallegro.

Presidente, l'emendamento 6.201 spiega, nel suo testo semplice e chiaro, tutto ciò che avrebbe dovuto fare il Governo, cioè proporci un testo semplice e chiaro, che chiarisse la linea in termini di contenuto e di metodo. Vediamo il confronto tra i due testi. Il Governo dice, al comma 1

destina i propri utili prioritariamente allo svolgimento delle attività statutarie nei limiti di cui alla lettera *d)*, adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti (...) e quindi rientra

così definite: «Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale (...)». Poi, però, queste attività di interesse generale vengono definite dell'articolo 4, «Al periodico aggiornamento delle attività di interesse generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta (...)». Quindi noi abbiamo delle finalità che vengono messe davanti come paravento, come cavallo di Troia, ma, poi, nelle modalità, il lucro è previsto e il potenziale il potenziale ampliamento o restrizione delle attività che possono essere ricomprese in questo ambito viene lasciato alla discrezionalità del Governo. Noi abbiamo proposto un testo alternativo, che vado a leggere. Potete valutarlo voi e non credo sia neanche importante o necessario spiegarlo. Dal nostro punto di vista, l'impresa sociale, cioè quella che svolge una funzione sociale, in sussidiarietà rispetto all'amministrazione pubblica, è un'organizzazione così definita: un «operatore dell'economia sociale il cui obiettivo principale è quello di avere un'incidenza sociale,» - quindi un impatto «piuttosto che ricavare profitto per i suoi proprietari o azionisti», che non è nemmeno del tutto escluso. Si precisa inoltre che: «Essa opera fornendo beni e servizi per il mercato in modo imprenditoriale e innovativo e impiega i propri profitti esclusivamente per perseguire obiettivi sociali». Non per altro, non per remunerare capitali, distribuire dividendi o, peggio ancora, per garantire proprio i personaggi che il senatore D'Anna ricordava: politici o coniugi coniugi di politici, poltrone riccamente compensate, mettendo nella loro disponibilità addirittura la possibilità di finanziare, a titolo personale a quel punto (ma da dove arrivano quei soldi lo sappiamo), questo o quel partito, questa o quella corrente, questa o quella fondazione. Non è stato possibile sopprimere l'articolo, ma lo si vuole migliorare o no? Infatti, tutto quello che non compare in una legge delega il Governo non lo può fare. Ma tutto quello che noi non precisiamo in termini di criteri prescrittivi, il Governo lo potrà fare,

Signora Presidente, questo emendamento introduce una materia che sarà affrontata con maggiore puntualità negli emendamenti successivi, ovvero la destinazione degli utili. A mio giudizio, il senatore Luigi Marino, nel dire che il testo proposto dalla Commissione del Senato è migliorato rispetto a quello della Camera, ha omesso di valutare che il testo del Senato riporta del Senato riporta in maniera più precisa il fatto che la destinazione degli utili non sia esclusivamente dedicata agli scopi di utilità sociale, cosa che invece si poteva leggere meglio nel testo della Camera. Quindi, l'emendamento 6.201, nella sua parte finale e al di là della parte iniziale, specifica che le imprese cosiddette sociali - poi vedremo perché è impossibile nel nostro ordinamento introdurre questa figura impiegano i propri profitti esclusivamente per perseguire obiettivi sociali. Sta tutto nella fumosità assoluta del termine «sociale». Tutta questa discrezionalità così ampia e incredibile è lasciata ad un Governo, che tra l'altro la deve ancora codificare attraverso i decreti delegati; quindi con un doppio livello di indeterminatezza - quello della norma e quello della norma in quanto delega che ci conduce a ritenere questo articolo 6 veramente inaccettabile e a ribadire la nostra assoluta contrarietà cercando di migliorarne il contenuto, almeno intervenendo sui principi della delega. In tal senso, devo ricordare a me stesso e a tutti i colleghi che siamo in fase di conferimento di delega, e non possiamo non essere precisi, come la Costituzione vuole, nell'indicare i principi cui il Governo deve attenersi nella stesura dei decreti delegati. Quindi, dire «prioritariamente» significa introdurre un elemento di incertezza che va da un 51 per cento fino ad un 99 per cento nella decisione che il Governo dovrà assumere su quanti degli utili debbano essere obbligatoriamente reinvestiti nell'attività sociale e quanti invece possano andare ai promotori e ai gestori dell'impresa. È quindi assolutamente indispensabile,

il male minore in quanto il male assoluto sta nell'articolo 6, cioè nella previsione che vi possano essere imprese private che possono gestire i loro bilanci, le loro attività, e quindi anche la loro presenza sul mercato, in maniera diversa tra loro perché qualcuna ha la qualifica di impresa sociale e altre invece hanno solamente la qualifica di impresa privata.

- adozione delle norme nella nostra legislazione. Credo quindi veramente che si debba riflettere su questo aspetto. La forzatura che già l'articolo 6 pone della differenziazione - quindi incostituzionale di per sé a monte - tra imprese, a seconda della qualifica che esse abbiano (sociali o meno), viene ulteriormente aggravata dal fatto che le imprese sociali possono anche essere imprese private fino ad un 49 per cento di ridistribuzione e di assegnazione degli utili. Mi sembra veramente aberrante;

6.202, perché in pratica questo emendamento prevede l'inserimento di alcune precisazioni. modificazioni: a) dopo le parole: "che svolge attività d'impresa" inserire la seguente: "esclusivamente"». Se andiamo a vedere la portata normativa che va a creare questo inserimento, possiamo notare che esso precisa in maniera particolareggiata qual è

una tipologia d'impresa completamente diversa; quindi la locuzione «esclusivamente» va a precisare questa

che fa tutt'altro lavoro sia esclusa e, per escluderla, c'è bisogno di inserire la locuzione «esclusivamente».

della destinazione degli utili. La parola «prioritariamente» sappiamo benissimo che è aleatoria; quindi ci vuole

dobbiamo fare in modo che questi utili vengano solo solo ed esclusivamente investiti per lo svolgimento delle attività statutarie. Altrimenti ci troviamo di fronte non ad un'impresa sociale, ma ad un'impresa punto e basta. Quindi, come diceva anche qualche altro collega, tutto ciò è tale da minare il principio della concorrenza e del libero mercato, perché di fronte a situazioni oggettivamente identiche si

Presidente, vorrei intervenire per sostenere questo emendamento, perché troppo a lungo e troppo spesso abbiamo discusso in quest'Aula della poca chiarezza dell'articolo 6.

Nel mercato, ahimè, troppo spesso ci si confronta con delle imprese sociali, perlomeno nella loro forma estetica, che poi nel loro corpo, nel loro agire e nel loro essere sono di fatto delle imprese commerciali, ma hanno trattamenti a volte troppo diversificati. Poco prima, soltanto un'ora fa, abbiamo votato un emendamento dove non si è voluto che l'Agenzia delle entrate operasse un maggior controllo su queste imprese sociali, adesso se vogliamo definire in maniera chiara e netta uno spartiacque tra i due mondi, per l'amor del cielo entrambi con ragioni di essere e di potersi